la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta.

2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio

n. 132, re- cante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e ver- samenti fiscali

e versamenti fiscali. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia nel testo approvato dalla Commissione, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, non appena pervenuto il parere della 5[a] Commissione. La prossima settimana, martedì 21 novembre, sarà discusso il decretolegge su misure contro il caro prezzi energia, approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia. Il calendario prevede inoltre la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione, nonché la discussione del disegno di legge per il contrasto della violenza sulle donne, approvato dalla Camera dei deputati. Per quest’ultimo procedimento la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito, all’unanimità, ai sensi dell’articolo 126, comma 12, del Regolamento, di autorizzare l’esame durante la sessione di bilancio. La seduta di mercoledì 22 novembre si concluderà alle ore 15, su richiesta di un Gruppo parlamentare. Giovedì 23 novembre, alle ore 15, avrà luogo il question time con la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il termine di presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12 di martedì 21 novembre. Il calendario della settimana potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge concernente la filiera tecnologico-professionale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Restano fermi gli argomenti previsti per le settimane dal 28 al 30 novembre e dal 4 al 7 dicembre. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito, all’unanimità, ai sensi dell’articolo 126, del Regolamento, di autorizzare, durante la sessione di bilancio, le Commissioni riunite 2[a] e 10[a] a discutere il disegno di legge, in sede referente, sull’oblio oncologico e la 7[a] Commissione a discutere il disegno di legge, in sede deliberante, sull’istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all’articolo 7-quater, del comma 3 con il seguente: “3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l’aeroporto dell’isola d’Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l’isola d’Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.” Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà. Signor Presi- dente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5[a ] Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull’approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 132, nel testo definito dalla 6[a] Commissione, modificato in conformità alla condizione posta dalla 5[a ]Commissione e accettata

di sottolineare che non c’è un elemento di novità nel fatto che il Parlamento costantemente ratifichi decisioni del Consiglio dei ministri tramite decreti-legge sui quali poi viene posta la questione di fiducia in questo modo, si snaturi il rapporto costituzionale tra potere legislativo e potere esecutivo. Dico che non è una novità perché questa cosa va avanti da molti, molti anni e da molti, molti Governi, di cui personalmente ho anche fatto parte. L’elemento quindi non è questo,

identico (due emendamenti identici, quindi: uno è già esistente nel fascicolo e il Governo, attraverso il relatore, ne fa presentare un altro identico). Perché? Perché c’è la necessità di segnalare la distinzione tra le forze politiche di maggioranza. Questo è il vero elemento politico

del Governo e del Parlamento italiano. Il vero elemento di novità è che una maggioranza che fa finta di essere unita su tutto, in realtà, è divisa su tutto. (Applausi). BOCCIA

di un’intesa nel Governo rispettosa dei tempi che quest’Assemblea aveva più volte spostato in avanti

ognuno di noi saprà di cosa sarà responsabile nel dibattito politico dei prossimi giorni - della discussione sulla proroga del mercato tutelato per fornitura di energia elettrica e gas. Stiamo cancellando

stiamo cancellando le risorse per gli enti locali; stiamo cancellando le risorse per gli ecobonus; stiamo cancellando la riorganizzazione di Aifa, ma - guarda caso - eravate disposti a tenere in vita le assunzioni per Consob. Ora, signor Presidente, non so quale fosse il meccanismo che avevate deciso di utilizzare per stabilire le priorità, ma quello che è evidente è che ad un certo punto avete trascinato i lavori oltre i termini, salvo poi impantanarvi,

Perché avete consentito a quel 10 per cento che non vuole la fatturazione elettronica di essere rappresentato da tutta la maggioranza in Parlamento? (Applausi). È proprio questo che avete fatto: avete preso in ostaggio i problemi reali del Paese per fare sponda a problemi che in realtà

ricordando a tutti che c’era una grande novità, finalmente un Governo politico coeso che non avrebbe più avuto le difficoltà con le quali, invece, si sono inevitabilmente confrontati gli Esecutivi degli anni passati, che, come sappiamo, avevano una base parlamentare molto più ampia. La verità è che questa ennesima fiducia dimostra quello che sta accadendo in queste settimane. Diciamocela tutta: o trovate una merce di scambio politica,

e l’altro elettorato vengono sufficientemente soddisfatti e in qualche maniera ingoiano il resto; oppure, quando non siete nelle condizioni di mettere in campo un elemento di scambio politico, ponete la questione di fiducia. come si vede, indipendentemente dai larghi numeri parlamentari, la maggioranza è molto meno coesa di come sembra, è molto più divisa di come sembra, è obbligata a ricorrere alla fiducia per nascondere questo elemento di divisione e lo fa anche in questo caso, non ci giriamo intorno. Infatti, nel momento in cui avete deciso, anche in questo caso segnando un elemento di assoluta novità, l’umiliazione del Parlamento e delle forze di maggioranza, decidendo che non possono nemmeno presentare emendamenti al disegno di legge di bilancio, segnando una clamorosa novità nella storia politica di questo Paese, ovviamente spostate spostate gli emendamenti da altre parti per cercare qualche forma di composizione, ma poi, come si vede, non vi riesce. Mi sembra infatti che quanto sta accadendo in queste ore testimoni davvero una profonda incapacità di governare questo Paese, che invece meriterebbe

si evidenzia che il Governo attuale ricorre esageratamente al voto di fiducia, anche perché io ho l’onestà intellettuale di ricordare che ho fatto parte della maggioranza di Governi che hanno fatto ricorso al voto di fiducia tanto quanto quello attuale. Tuttavia - devo dire la verità - sono quasi contenta di vedere che lo stato comatoso dell’attuale maggioranza sia già conclamato dopo solo un anno di governo. Lo spettacolo a cui abbiamo assistito oggi, colleghi, va oltre il fatto che voi ricorriate al voto di fiducia, com’è naturale che sia; il fatto è che voi siete arrivati al voto di fiducia dopo liti

mi spiace che abbiate contratto la discussione, mi spiace che il Parlamento sia stato schiaffeggiato da un atteggiamento tutto

Questo emendamento era una risposta immediata e forte a una mancanza che il Governo aveva avuto di recente, ma con il voto di fiducia oggi di fatto dobbiamo rinunciare a dare

ordinatamente e costruttivamente, eravamo riusciti a fare in Commissione e che purtroppo trova un epilogo che possiamo definire un po’ indegno. Questo è doveroso ricordarlo. In questo provvedimento ci sono articoli condivisibili perché dettati da mere ragioni di buonsenso, ma ce ne sono altri che non dovrebbero stare in un proroga termini, poiché trattano questioni che meritano un riordino generale e ce ne sono altri ancora che riflettono il profilo regressivo in materia fiscale del Governo. La norma sulle criptovalute, a prescindere dalla scadenza, è uno scudo fiscale su una forma di transazione finanziaria adoperata anche dalle organizzazioni criminali internazionali per attività di riciclaggio e finanziamento del territorio e non è un caso che la Commissione europea abbia

Vogliamo nuovamente ribadire la nostra contrarietà al concordato preventivo biennale previsto dalla legge delega in un Paese dove il 13 per cento dei contribuenti versa il 62 per L’idea che lo Stato negozi con i soggetti che hanno eluso il fisco una specie di amnistia è la negazione di qualsiasi principio di uguaglianza fiscale e di giustizia sostanziale. Allo stesso tempo, non si comprende la ratio alla base di alcuni articoli con un vero e proprio rischio di eterogenesi dei fini. È il caso dell’articolo 7, che anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre il termine di utilizzabilità dei crediti d’imposta per il contrasto al caro energia delle imprese. Lo ha denunciato Confesercenti durante le audizioni in Commissione: considerando che tali crediti possono essere ceduti, è evidente che con l’anticipo molte delle imprese possano trovarsi nella situazione di incapienza da compensazione. È il caso dell’articolo 15 in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato d’insolvenza. La proroga di ulteriori per il completamento della cessione dei complessi aziendali non tiene conto dei creditori che rischiano quindi di veder pregiudicata la loro posizione. Meritava invece un ragionamento strutturale la norma sul lavoro agile; se la proroga indubbiamente risponde all’esigenza reale di una parte del mondo del lavoro, proprio per questo occorre superare la logica emergenziale, individuando uno specifico fondo che permetta di ricorrere al lavoro agile sulla base di specifiche esigenze e i cui eventuali risparmi potrebbero essere adoperati per altre finalità. Insomma, Presidente, c’è da essere preoccupati per le modalità con cui il Governo si sta muovendo sui temi economici, la frammentarietà delle misure, la tendenza a rinviare i problemi, la mancanza di una logica programmatoria, l’assenza di una politica per lo sviluppo e la crescita economica. Tutti gli attori interpellati in questi giorni sulla legge di bilancio fotografano questo quadro; lo fa l’Ufficio parlamentare di bilancio, denunciando la mancanza di programmazione, l’incertezza delle risorse o la loro inadeguatezza per alcune delle misure annunciate, lo fanno i sindacati che denunciano la mancanza di misure per restituire potere d’acquisto ai lavoratori e ai pensionati e lo fa Confindustria che lamenta assenza di misure a sostegno degli investimenti privati e soprattutto di una strategia finalizzata alla crescita e alla competitività. Presidente, non basta dire infatti che le risorse sono poche e che il quadro internazionale è difficile per giustificare una simile politica economica. Le risorse si reperiscono contrastando l’evasione fiscale, uscendo dalla logica pilatesca dei tagli lineari, mettendo in campo politiche che facciano da moltiplicatore economico, sfruttando appieno il PNRR. Le risorse si reperiscono assumendo scelte politiche e non assecondando bisogni elettorali che sono quelli che fino ad ora hanno guidato l’Esecutivo, si tratti della riforma fiscale, della legge di bilancio e anche di questo provvedimento.

che sarebbe valsa comunque, a prescindere dalla fiducia; noi siamo di fronte all’emanazione di un decreto-legge proroga termini di fatto a pochissimi mesi dal precedente. Quello che quindi aggiungo alle considerazioni fatte prima è che non solo non vedo una grande lucidità nella gestione politica, ma colgo anche una decisa improvvisazione nel mettere a fuoco e in linea i temi. È chiaro infatti che un provvedimento di questo genere, a così breve distanza dall’altro,

sono l’anticipo termini per utilizzare i crediti di imposta, elementi riconducibili alla questione del lavoro agile, l’ennesima proroga sulla questione degli organi Aifa Aifa e tutte le questioni legate al pagamento delle supplenze dei precari della scuola. Ci sono inoltre le attività emergenziali sulla crisi in Ucraina

vicende come queste, una forza politica responsabile, non ideologica e non necessariamente contro come la nostra, che valuta singolarmente proposta per proposta, in un quadro di fedele opposizione con la capacità di guardare agli interessi del Paese (stiamo parlando magari di un metodo che non è eccezionale, ma comunque di in alcuni casi possono addirittura dare una mano a situazioni di difficoltà), avrebbe avuto un atteggiamento laico. Tanto più che avevamo in mente, in questo provvedimento, di farci carico della questione cui accennavo prima e che voglio riprendere, perché, quella sì, per noi è una priorità assoluta. Nel 2021 Luana D’Orazio è morta schiacciata da un macchinario solo pochi giorni fa, il 14 novembre, un’altra lavoratrice, Anila, di ventisei anni, è morta schiacciata da un macchinario. macchinario. (Brusio). Scusate, colleghi, capisco che il tema possa non interessare, ma a me sembra abbastanza singolare che voi chiacchieriate di fronte a questi argomenti. Io penso che si debba necessariamente fare il punto su quello che è accaduto. Lo dicevo prima e lo dico ora più puntualmente.

prevedeva che i datori di lavoro mettessero una sorta di dispositivo di blocco su quei macchinari che potevano ingenerare situazioni come queste. Di fronte a questo parere positivo, eravamo tutti molto soddisfatti e molto contenti di aver potuto contribuire a una piccola cosa utile nel Paese.

io capisco perfettamente che, per cercare di creare un positivo sistema di aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, bisogna incentivare il cambiamento dei macchinari e quindi magari farsi carico di provvedimenti economici a sostegno. Lo faremo nella legge di bilancio,

avesse potuto valutare l’appropriatezza dei provvedimenti, in uno schema libero da ideologismi, provando magari a migliorare questo atto, con un intervento ulteriore, però tanto importante per dare la sensazione che la politica guarda a quello che accade nel Paese, se ne fa carico con grande senso di responsabilità e prova a trovare delle soluzioni, anche quando le questioni sono complesse. Naturalmente, quando parlo di questi temi, ne parlo sapendo che in quest’Aula ci sono delle persone che più di me hanno sensibilità e competenza (penso ad Annamaria Furlan e alla senatrice Camusso). Quindi c’è la massima disponibilità a unire le forze e a lavorare perché un intervento sia il più possibile completo. Però questa libertà di movimento, che è mancata nella decisione del decreto attuale, non ci consente di fare quell’intervento e non ci consente nemmeno di giudicare singolarmente le questioni, senza pregiudizio e senza ideologia,

perché avete evidenziato che i problemi li avete e sono piuttosto seri; al Paese, perché non avete consentito che venisse inserita oggi una norma sensata, che sarebbe stata tempestiva rispetto a quello che è accaduto nei giorni scorsi, considerati il dolore di quella famiglia e quello di tutti quei lavoratori che sono incorsi in incidenti nei luoghi di lavoro. In più, non ci avete nemmeno consentito di valutare in maniera il più possibile spassionata le singole voci dentro un decreto-legge omnibus di proroga termini. A proposito

di un Paese in una morsa anche in questo caso ideologica: da una parte, un sindacato che si schiera contro una manovra ancor prima di conoscerla; dall’altra parte, un Ministro che pensa di affrontare con il pugno duro ogni questione, lasciando invece del tutto

pubblico in qualsiasi sede. Siccome è evidente che non siete in grado di produrre meccanismi di semplificazione e di miglioramento della parte autorizzativa, e che state bloccando l’economia e i trasporti in questo Paese,

una metropolitana, oppure che potessero andare al lavoro in sicurezza, che è un bisogno primario, essenziale e inalienabile delle persone che lavorano. Siamo invece costretti a vedere lo spettacolo di una maggioranza che, siccome non sa se prenderà il treno questa sera, perché domani non è certo che con lo sciopero ci saranno i treni, mette la fiducia su un provvedimento. Glielo dico sinceramente, signor Presidente: a me cadono le braccia,

quello fiscale e la legge di bilancio, sostanzialmente doveva affrontare alcune questioni, a partire dal fatto che si parla di proroghe

cittadini, giovani, precari, famiglie, in particolare con un basso reddito. Per esempio, su tutto il sistema della casa e degli affitti, niente è stato affrontato e niente verrà affrontato, perché nei provvedimenti in corso non c’è una risposta alla questione degli

Il punto è che bisogna costruire un messaggio di fiducia perché qualcuno si impegni. Ad esempio, oltre a non avere alcuna politica sulla questione della casa

in nessuno di questi provvedimenti c’è una risposta a questo dato della precarietà. La precarietà è la certezza. E precarietà vuol dire bassi salari e un basso introito. un basso introito. Non basta pensare che si può dare una risposta parziale e temporanea con il cuneo fiscale. Io insisto sul problema dei salari, sul problema delle retribuzioni, sul fatto che c’è una povertà economica di migliaia, milioni di persone,

la questione della stabilità. Qui, addirittura, siamo all’assurdo. Noi lasciamo andar via delle persone che, assunte

Le nostre intelligenze se ne vanno. Perché non restano in Italia? Perché non hanno nessuna possibilità per il futuro. Se hanno bassi salari e precarietà,

Francamente, in questi mesi, piano piano, sono stati smantellati tutti i momenti di concertazione, coinvolgimento e coesione, per far partecipare, ad esempio, le autonomie locali e i Comuni.

queste settimane, abbiamo stabilito un modus operandi che ha portato a un miglioramento del testo che è approdato oggi in Aula. È stato svolto un lavoro emendativo importante, che ha lasciato spazio a tutte le forze politiche. Per questo va ringraziato anche il Governo, che ha seguito un lungo confronto in Commissione. L’altro aspetto di cui mi preme parlare, però, è quello del merito e su questo credo che Forza Italia abbia fatto un lavoro importante, consentendo al decreto-legge di essere licenziato oggi qui in Senato in una versione migliore e soprattutto più incisiva. La Commissione finanze, durante il suo esame, ha inoltre introdotto ulteriori modifiche di iniziativa parlamentare: ne cito solo alcune d’iniziativa dei senatori del Gruppo di Forza Italia. La Commissione finanze ha approvato, su nostra iniziativa, una proroga per i contratti di locazione delle unità immobiliari in regime di edilizia agevolata ai militari e agli uomini delle Forze di polizia, consentendo loro la prelazione sull’acquisto quando gli immobili vengono posti sul mercato. C’era il rischio che questi servitori dello Stato venissero cacciati dalle abitazioni nelle quali vivono da molti anni. Un altro tema è quello della formazione di chi si impegna nel salvamento in acqua dei bagnanti, per individuare i soggetti più adatti a fornire la più opportuna formazione. Servivano norme per dare maggiore certezza a questo percorso percorso di formazione e le abbiamo introdotte. È un lavoro importantissimo quello di salvare vite in pericolo, che non si può lasciare sicuramente all’improvvisazione. Vorrei poi ricordare la norma che consente la migrazione di dati della pubblica amministrazione sul cloud nel tempo necessario a completare queste operazioni, per renderla di una norma fondamentale per queste aziende aziende energivore, in un momento in cui i prezzi dei prodotti energetici sono ai massimi livelli per un comparto che è il motore del settore delle costruzioni e che contribuisce a una larga parte del PIL italiano. In Commissione finanze abbiamo poi introdotto una norma che ci è stata chiesta dai Comuni, che riguarda la semplificazione del prospetto delle aliquote IMU e con essa anche la proroga della revisione della spesa dei Comuni che necessitano di più tempo per individuare il complesso delle spese da razionalizzare. Resta fermo che non verrà toccata né la spesa per i diritti sociali, né le politiche sociali e la famiglia. Nel testo del decreto-legge il Governo ha individuato innanzitutto la necessità di prorogare fino alla fine dell’anno la misura del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa sulla quota capitale dei mutui destinati alle giovani coppie fino a trentacinque anni e ad altri soggetti fragili. È un provvedimento che ha funzionato, posto che nel primo semestre di quest’anno hanno usufruito di questa possibilità quasi 35.000 mutuatari. Gli stanziamenti sul Fondo sono pari a 505 milioni nel 2023; si stimano acquisti di immobili per circa 12 miliardi di euro, posto che le garanzie

Sono quindi stati rimessi in termine fino a ottobre tutti coloro che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia a luglio di quest’anno, non erano riusciti ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per le assicurazioni obbligatorie che erano in scadenza, come ricorderete, a fine luglio. prorogati anche i termini delle condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali per le cessioni e assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. È stato differito il termine che ora consentirà, in caso di variazione dell’IBAN, l’accredito dell’indennizzo del fondo indennizzo risparmiatori (FIR), spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, come ampiamente illustrato in discussione generale dal senatore Zanettin. Inoltre, i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno adempiere agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente entro un termine più congruo. di utilizzabilità dei crediti d’imposta destinati a contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas sostenuti dalle imprese in questo primo semestre 2023. prorogato il termine per completare il programma di cessione di complessi aziendali nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza. pur nella varietà delle norme in esso contenute, il decretolegge contiene tante disposizioni che consentiranno alla macchina pubblica di funzionare meglio a favore dei cittadini e consentirà alle imprese di operare meglio nei propri settori economici. Come ho già detto (ma intendo in questo momento ribadirlo) molte modifiche sono state proposte proprio dai senatori del Gruppo Forza Italia, che hanno lavorato in perfetto accordo con il Governo. Per questa ragione annuncio il voto convintamente favorevole dei senatori di Forza Italia sulla fiducia posta dal Governo sul provvedimento in

innanzitutto ringraziare il vice presidente Melchiorre, la relatrice Zedda, tutti i componenti della Commissione e anche il

Volevo quindi ringraziare a questo punto sia la Commissione che il Governo per aver accolto anche gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. Ne vorrei ricordare alcuni.

fiducia che il Governo ha posto su questo provvedimento, si impedisce innanzitutto al Senato e quindi al Parlamento di migliorare ancora il provvedimento che quindi, nella sua complessità, risulta non sufficiente e non idoneo a risolvere i problemi dei cittadini e soprattutto delle imprese. Questo è l’ennesimo provvedimento d’urgenza che manca di una visione e di un sistema di soluzioni al problema economico e al problema sociale del Paese. Si tratta inoltre di anticipa la legge di bilancio, quello che avverrà poi nella prossima manovra, perché questo provvedimento, che nasce come decreto proroghe normative e versamenti fiscali, si trasforma in un vero e proprio decreto

di governo, perché di fronte ad un Paese che ormai è in stagnazione, con una produzione industriale che a settembre è crollata del 2 per cento, con consumi che sono crollati, una crescita economica che è partita da uno zero virgola ma sempre più sta perdendo la virgola e si avvicina allo zero, il Governo festeggia il giudizio stabile di alcune società di rating. Vorrei, però, ricordare che il giudizio stabile lo abbiamo sempre avuto, almeno negli ultimi anni, dopo il giudizio stabile c’è il precipizio, per cui non ci sarebbe nulla da festeggiare. (Applausi). Forse ciò che andrebbe festeggiato è che se le società di rating hanno dato questo giudizio stabile sui conti pubblici, significa che non esiste nessun buco di bilancio paventato dal Governo e da molti Ministri. Allo stesso tempo, finalmente anche il ministro Giorgetti ha tolto la maschera, perché proprio ieri in audizione

condividiamo e cioè che la prossima legge di bilancio sarà invece espansiva nei confronti dei lavoratori. Peccato però che i lavoratori protesteranno, nei prossimi giorni e settimane, in tutte le piazze d’Italia. Peccato anche che l’OCSE

Detto questo, entrando nel vivo del provvedimento, io l’ho definito un “decreto tagli, tasse e e favori agli evasori”. Cercherò a questo punto di dimostrarvi quanto da me evidenziato. Sul fronte casa

non prorogate l’aliquota al 21 per cento e nella legge di bilancio portate l’aliquota sugli affitti brevi al 26

in relazione anche all’introduzione della fatturazione elettronica, dall’8 all’11 per cento. Questa misura sulle ritenute fiscali e sui bonifici parlanti era stata introdotta per contrastare l’evasione fiscale nel campo dell’edilizia prima dell’introduzione della fatturazione elettronica. Oggi, con questa misura di aumento della ritenuta fiscale, andate a compromettere la liquidità di migliaia di imprese edili che vedranno ridotte le loro entrate commerciali. Non confermate poi l’imposta sul valore degli immobili all’estero; anzi, aumentate, anche qui, l’imposta dallo 0,76 per cento. Non prorogate l’agevolazione sulla detrazione IVA per gli acquisti di immobili di classe A e B, tagliate i bonus mobili, portandoli da 8.000 a 5.000 euro, non rinnovate il potenziamento del fondo per la sospensione delle rate dei mutui. Sulla casa però non finisce qui. Il senatore Lotito parlava di grande successo del Governo e della maggioranza con riferimento ai giovani, agli under trentasei, sul rinnovo e sulla proroga del fondo di garanzia dell’80 per cento. Attenzione; la maggioranza e il Governo hanno dimenticato di rinnovare le agevolazioni sulle imposte di registro, sulle imposte ipotecarie e su quelle catastali. Sono tali agevolazioni che hanno permesso ai giovani di acquistare gli immobili e non solo la garanzia sull’immobile. Presidente Lotito, sa quanto viene a costare in più acquistare una casa per un giovane under trentasei del valore di 250.000 euro? Più 10.250 euro. State andando a mettere le mani nelle tasche dei giovani. Sul fronte famiglia non rinnovate lo sconto sulle accise del carburante, non confermate l’IVA ridotta del 5 per cento sui prodotti dell’igiene intima e dell’infanzia, e dell’infanzia, riportandola al 10 e al 22 per cento. Mettete le mani nei portafogli delle donne; una vergogna. Sempre sul fronte famiglia, non rinnovate il mercato protetto per quanto riguarda il bonus sociale energia; attenzione, altri Paesi europei hanno ricevuto la proroga da parte della Commissione europea in tempi molto ristretti. Sono mesi che andate a interloquire con l’Europa e l’Europa non vi sta dando l’autorizzazione. Questo dimostra la vostra incapacità e la vostra non credibilità a livello internazionale.

Sul fronte imprese, c’è innanzitutto la mancata proroga del superbonus 110 per cento, che avete sostenuto in campagna elettorale e adesso infangato con una falsa narrazione (altro che buco di bilancio). Dopodiché non andate a prorogare l’ACE, l’aiuto alla crescita delle imprese, e sottraete al mondo delle imprese oltre 4,5 miliardi. Non rinnovate i crediti d’imposta su formazione, ricerca e transizione 4.0; nello stesso tempo, il concordato preventivo biennale, che avete sbandierato quale misura contro l’evasione fiscale, sapete a chi sarà applicato? Ai contribuenti affidabili, a quelli che hanno un indicatore ISA superiore all’8 per cento, ovvero a chi già paga le tasse. Sarebbe forse stato più opportuno andare ad applicare questo strumento, che avete definito anti-inflazione, agli inaffidabili per il fisco e non agli affidabili. Sul fronte evasione c’è l’ennesima sanatoria per gli evasori cosiddetti digitali, cioè per coloro che hanno realizzato plusvalenze dalle criptovalute e - ahimè - hanno dimenticato di dichiararle e di pagare le tasse.

in tema di ristrettezza mentale e di mancanza di visione: «Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che è oltre la loro portata».

il Governo fa un passo avanti importante nella giusta direzione, per rispondere alle istanze di famiglie e aziende, che in questi anni stanno affrontando sfide enormi, conseguenti prima alla pandemia e poi alla crisi innescata dai conflitti in corso, ma anche dai cambiamenti climatici e soprattutto dall’inflazione. Il decreto-legge in questione si compone di 17 articoli e contiene numerose proroghe di termini normativi e versamenti fiscali. L’obiettivo è quello di alleviare parzialmente la pressione fiscale sui cittadini, diluendo i termini dei versamenti ed ampliando invece le tempistiche a disposizione per usufruire di facilitazioni e garanzie. Come accade in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione, per cui è previsto lo slittamento al 31 dicembre (prima era il 30 giugno) dell’estensione della garanzia massima all’80 per cento a valere sul fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, con specifici requisiti di reddito ed età (i giovani di età non superiore ai trentasei anni e le giovani coppie con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui). Il fondo di garanzia è uno strumento importante, che ha ricadute sia sulle famiglie, sia sul settore dell’edilizia (parliamo sempre di famiglie e di imprese). Un occhio di riguardo è stato riservato anche a chi, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non ha potuto effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza dal 4 al 31 luglio; versamenti che, con la proroga, saranno considerati tempestivi anche se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023. Il provvedimento prende anche in considerazione le società. In questo ambito viene prorogato al 30 novembre il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni non strumentali ai soci e quelle di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, viene anche prevista la rimodulazione del versamento dell’imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, sempre entro il 30 novembre 2023. Sempre per andare incontro alle esigenze delle categorie più fragili, viene prorogato lo smart working per questi soggetti, che potranno usufruirne per tre mesi in più, fino al 31 dicembre Novembre 2023 30 settembre). Un’altra proroga riguarda un altro ambito importante della nostra società, ossia il mondo della scuola: viene infatti autorizzata fino al 31 dicembre la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Nel corso dell’iter sono stati numerosi gli interventi emendativi da parte di tutti i Gruppi.

La parte più importante è quella relativa alle infrastrutture digitali, l’acquisto di beni e servizi strumentale alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la digitalizzazione dei provvedimenti. A tal proposito, ricordo l’emendamento in modifica al decreto-legge del 24 febbraio 2023, è fondamentale, nel caso del Piano di ripresa e resilienza, spendere bene le risorse e utilizzare questo strumento per allenarsi a operare e ad agire in modo programmatico e attento sul tema degli aiuti di Stato, operando in modo preventivo. Altro argomento importante è il fondo di solidarietà comunale. A questo proposito, grazie anche a un nostro emendamento, è stato prorogato al 30 ottobre il termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardante le risorse integrative assegnate nel 2022, a fronte dell’obbligo di raggiungimento di determinati risultati. Tra i temi affrontati, vi è anche quello - sembra vecchio nel tempo, ma è sempre attuale - delle quote latte, che ci sta a cuore perché tocca molte aziende del settore dell’allevamento che, oltre alle difficoltà dovute alla crisi, in questi mesi sono costrette anche a sostenere il peso dei rimborsi. Nelle campagne, nei periodi compresi tra il 1995 e il 1996, e tra il 2008 e il 2009, l’Italia avrebbe infatti applicato regole di compensazione non corrette rispetto a quanto previsto dai regolamenti comunitari, fissando criteri di priorità nell’attribuzione delle quote inutilizzate, non in linea con tre sentenze della Corte di giustizia europea. L’emendamento approvato prevede la riapertura dei termini di accesso alle misure di rateizzazione dei debiti. La proposta si inserisce nel percorso già avviato per chiudere in parte la vicenda. Sulla programmazione regionale interviene, anche qui, un emendamento proposto dal nostro Gruppo, che prevede che, in attesa dell’approvazione della riforma del quadro di governance dell’Unione europea, si possa lavorare a basso rischio per quanto riguarda i termini in essere. Abbiamo poi portato avanti l’emendamento cui viene individuata l’entrata in vigore del divieto a partire dal terzo mese successivo a quello dell’approvazione di un sistema di certificazione a basso rischio, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. In tal modo vogliamo tutelare una filiera importante per il settore economico ed energetico del Paese, mantenendo comunque alta l’attenzione alla tutela ambientale, evitando nell’immediato di alimentare ulteriormente la crisi energetica in cui versa il Paese.

occorre intervenire con ogni strumento a disposizione per sostenere le famiglie e le imprese a basso reddito, i ceti medi, nonché il mondo del lavoro, al fine di garantire l’occupazione e di far crescere l’economia e il benessere generale. Un passo alla volta, la Lega e il Governo portano avanti un programma per supportare famiglie, imprenditori, artigiani, commercianti, partita IVA, e per rendere l’Italia un Paese più moderno e sicuro, a misura di famiglia, con al centro il lavoro. Il fine ultimo della politica deve essere il bene del Paese e il benessere dei suoi cittadini: questo l’obiettivo che guida da sempre la nostra azione. C’è una frase, che io credo sia importante ricordare in questo Parlamento, di Luigi Einaudi, che deve ispirare l’azione nostra, l’azione del Governo: il denaro dei contribuenti deve essere sempre sacro. E con questo monito, io dichiaro, su questo importante provvedimento, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione. (Applausi).

Signor Presidente, credo che il sottosegretario Freni e il Governo possano testimoniare il fatto che il nostro Gruppo si era accostato con spirito costruttivo all’iter di questo provvedimento, nella consapevolezza che, insieme al decreto fiscale, che discuteremo a breve, esso costituisce l’ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell’anno, prima della legge di bilancio. Ed è proprio per gli evidenti limiti di quest’ultima, emersi anche durante le audizioni, e per le scelte nel merito e nel metodo che il Governo ha fatto nella presentazione della manovra, che provvedimenti come questo si sono caricati di aspettative e attese da parte degli enti locali, del mondo economico e delle imprese e dei cittadini ed evidentemente anche delle forze politiche, in primis quelle di maggioranza, che hanno caricato il provvedimento di tutte le attese tradite dei propri rispettivi elettorati. Siamo quindi arrivati alla non edificante rappresentazione di oggi, con le tensioni nemmeno troppo mascherate tra maggioranza e Governo, e poi al voto di fiducia. Dopo settimane di tentennamenti, fughe in avanti e marce indietro, sempre da parte della maggioranza, non solo le aspettative delle forze politiche, ma anche i reali bisogni di protezione sociale e di crescita economica, cui la legge di bilancio non corrisponde, vengono in grandissima parte disattesi, anche nel testo che oggi è arrivato in Aula, così come emendato dalla Commissione. Le richieste e le esigenze degli enti locali hanno trovato modestissima o nessuna accoglienza nel testo. Si continua a proseguire con un approccio che scarica sui Comuni costi e compiti, senza adeguate dotazioni finanziarie e senza nemmeno la flessibilità che l’ANCI ci aveva chiesto. Verrebbe da domandarsi a quale autonomia spesso facciano riferimento i colleghi della maggioranza, se poi i Comuni e gli enti locali vengono privati di ogni flessibilità. Purtroppo, non sono bastati a cambiare il segno generale dell’intervento i nostri emendamenti approvati in Commissione sull’utilizzo, per i Comuni, delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui o sulla relazione degli obiettivi di servizio. Ricordo, infatti, che a gravare sui Comuni permane ancora oggi il taglio lineare della spending review, contenuta in manovra, di 200 milioni di euro, cui si aggiungono gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale, che è cosa sacrosanta, ovviamente, per i dipendenti pubblici, ma che pesa per intero sui bilanci di questi enti. Non vi è nulla di significativo sul tema della casa, sui mutui, sul fondo affitto e prima casa, nonostante le trionfali dichiarazioni dei colleghi di maggioranza. Non è abbastanza, infatti, rispetto al tema emergenziale che, soprattutto nelle grandi città, è diventata la questione degli affitti o dell’acquisto della casa. Sulla questione della sanità sono già intervenuti dei colleghi, tra cui la collega Zampa ieri in discussione generale. Abbiamo trovato non accettabile l’approccio del Governo rispetto ad Aifa, l’importante agenzia del farmaco.

Signor Presidente, ringrazio lei e anche i colleghi, se avranno la cortesia di ascoltarci, così come noi abbiamo ascoltato loro. Stavo dicendo, a proposito delle terre alluvionate dell’Emilia-Romagna, che i nostri emendamenti, che andavano ad alleviare la situazione di imprese e cittadini, non sono stati accolti. Ciò che è stato accolto è ben poca cosa rispetto al bisogno e soprattutto rispetto alle promesse che il Governo, con la Presidente del Consiglio in testa, aveva fatto a quei cittadini e a quelle imprese. Noi continueremo a vigilare su questo. Il capitolo dell’energia è disastroso - com’è stato già riferito da altri colleghi - non tanto per quello che c’è nel testo, ma soprattutto per quello che non c’è, in una fase in cui il costo della bolletta erode salari e redditi, soprattutto per le fasce meno abbienti. Il sacrosanto principio europeo della libera concorrenza va difeso quando avvantaggia i consumatori ed è quello lo spirito con cui l’Europa si è accostata al tema del libero al tema del libero mercato per l’energia elettrica. Non è un caso - com’è stato ribadito - che altri Paesi europei nelle nostre stesse condizioni abbiano negoziato per tempo un differimento dell’entrata in vigore del libero mercato. Noi in questo provvedimento non riusciamo a fare nulla. So che era era previsto un ordine del giorno sul tema, che evidentemente non verrà discusso, poiché il Governo ha scelto di porre la fiducia sull’intero provvedimento. Mi risulta evidente e credo lo risulti anche a voi che il quadro complessivo del decreto-legge è alquanto striminzito nelle risorse messe a disposizione e rispetto alla visione generale di politica economica che il Governo prospetta.

per incrementare i consulenti e i collaboratori del Gabinetto del Ministro. (Applausi). A questo si aggiungono altre misure, sempre volte a incrementare la dotazione organica di quel Ministero nelle posizioni centrali e non sui territori, dove ci sarebbe, sì, bisogno di più ispettori e di più personale. Le ultime assunzioni stabilite sul tema della sicurezza sul lavoro sono frutto del lavoro del del Governo Draghi: gli ispettori che oggi sono entrati in funzione e stanno facendo la formazione derivano dalle scelte di un Governo precedente, questo mentre si chiede la proroga per la riorganizzazione dello stesso Ministero. In effetti, dopo che, prima dell’estate, era stata annunciata l’abolizione da parte della ministra Calderone, stentiamo a vedere quale disegno complessivo di revisione e riorganizzazione delle politiche attive del lavoro il Governo abbia in testa. E non basta una piattaforma tecnologica per risolvere un grave problema di carenza di manodopera e di disoccupazione giovanile. (Applausi). Signor Presidente, per queste e per molte altre ragioni, che sono state illustrate dai colleghi delle opposizioni prima di me, nel merito e soprattutto anche per il metodo con cui oggi si arriva all’ennesimo voto di fiducia, convintamente espongo e annuncio il voto contrario del Gruppo Partito Democratico.

il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è ancora una volta una risposta rapida ed efficace di un Governo che agisce e soprattutto sa come agire; un Governo che come obiettivo primario si pone la tutela dei cittadini, specialmente quelli più fragili; un Governo che ha compreso che il settore dell’impresa è non una miniera di diamanti da depredare senza scrupolo, bensì la pietra d’angolo che contribuisce a sorreggere con solidità l’economia della nostra Nazione (Applausi); che ha chiaro di dover essere promotore dell’impresa e suo collaboratore. Le disposizioni contenute nel testo legislativo in discussione identificano determinati termini normativi e versamenti fiscali e, considerando la tutela dei soggetti da essi interessati come prevalente rispetto alle relative entrate statali, offrono delle deroghe temporali essenziali affinché tale tutela possa aver luogo. Lo Stato, dunque, si presenta non come un inflessibile esattore, non come una specie di sceriffo di Nottingham pronto a prendere ai poveri per dare ai ricchi, ma come cooperatore e protettore (Applausi), al lavoro per il ripristino del rapporto di fiducia tra le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni, che da anni sono abbandonate da politiche tese ad altri interessi. Non intendo operare una nuova disamina del provvedimento articolo per articolo, già eseguita da altri colleghi e soprattutto in altre sedi.

che possa aiutare le categorie interessate considerate in situazione di fragilità a raggiungere il porto sicuro di una stabilità economica e familiare, qual è l’acquisto della prima casa. La prima casa, che qualcuno in quest’Aula ardentemente brama di tassare da anni, rappresenta un momento di respiro nella famiglia, nonché un diritto fondamentale che noi intendiamo e intenderemo sempre salvaguardare. Con questa misura di proroga, il Governo ribadisce l’idea che lo Stato c’è e sta dalla parte del cittadino, di chi è più fragile, di chi ha appena cominciato a progettare i propri piani di vita futura, desidera una famiglia e la desidera nella nostra Italia. Vorrei poi menzionare l’articolo 3. Anche questa disposizione individua una situazione di fragilità nella nostra terra e - vi piaccia o meno - eleva il sostegno ad essa a priorità nell’azione di Governo. La misura, così come uno degli ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo, si pone nell’insieme di provvedimenti a supporto dei territori colpiti dagli effetti dei terribili eventi meteorologici occorsi negli ultimi mesi. Contrariamente a quanto dichiarato da alcuni leader dell’opposizione, il Governo non si dimentica di loro ed è sempre al loro fianco in questa emergenza. Ancora, in tema di situazioni di fragilità, visto che in qualche intervento precedente si sono fatte narrazioni della realtà un po’ fantasiose, vorrei rammentare l’articolo 8 che proroga la possibilità per i lavoratori fragili di continuare a svolgere le proprie mansioni lavorative dalla postazione di propria preferenza. Il lavoro non può essere concepito come separato dalla dignità e per questo non deve mai rappresentare un rischio per la propria salute. La misura trova le proprie fondamenta su questa solida base. In questo delicato, delicatissimo momento storico, consentitemi però

senza mezzi termini. (Applausi). La condanna dell’invasore russo è radicata nella nostra memoria dai tempi dell’ottobre del 1956, in cui convintamente eravamo a fianco di migliaia di studenti, braccianti e operai che manifestavano contro la presenza sovietica in Ungheria. Questa è la nostra storia, una storia di coerenza, e nessuno può pensare di scalfirla. Con altrettanta sincerità oggi nelle piazze siamo accanto al popolo di Israele (Applausi), senza se senza gli imbarazzanti distinguo a cui oggi sono costretti quanti si propongono come testimoni dell’orrenda tragedia della Shoah, ma non si indignano di fronte agli slogan che inneggiano ad Hamas e scandiscono ritornelli di morte per lo Stato di Israele. Noi non abbiamo bisogno di veli o di paraventi, perché la coerenza è un valore, un vessillo e non una parvenza. Desidero infine sottolineare l’emendamento approvato in Commissione finanze che prevede la proroga della sospensione del meccanismo del payback per le aziende sanitarie. Si tratta di una misura essenziale a favore di un settore, qual è quello sanitario che, nel passato, è stato troppo spesso vittima di tagli indiscriminati e gli effetti di questi tagli li vediamo e li gestiamo noi oggi, purtroppo. STENOGRAFICO 16 Novembre 2023 nell’ottica di una cooperazione solidale ed efficiente a tutti i livelli dello Stato. Erano anni che questa misura poteva essere affrontata, ma lo deve fare questa maggioranza, quella del Governo delle idee che diventano azioni. azioni. Concludo con una riflessione che sembra necessario ribadire, visti gli interventi precedenti. Siamo gente di coerenza e di coraggio e il voto favorevole che il Gruppo Fratelli d’Italia si accinge a esprimere non è mai stato dato per scontato da questo Governo, ma è sempre stato condiviso e per questo ringrazio il Governo. Non sono mai ordini calati dall’alto su cui, per eseguire la linea imposta dal partito, non è consentito parlare. Questo accadrà forse altrove, in qualche piattaforma finta, ma non accade in Fratelli d’Italia. La storia di Fratelli d’Italia è una storia libera di persone che lavorano in condivisione per un obiettivo comune ed unitario, il bene dell’Italia. Per tutte le ragioni anzidette, il Gruppo Fratelli d’Italia, che in questo momento rappresento, come già anticipato, annuncia il suo voto favorevole.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

i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l’appello nominale.

Licheri Ettore Antonio C Licheri Sabrina

Sto andando più veloce che posso, Presidente. PRESIDENTE. Proseguiamo con i tempi consueti e normali.

Anna Politkovskaja era una giornalista russa in prima linea nella difesa dei diritti umani. Lavorava alla «Novaja Gazeta», venne assassinata diciassette anni fa per farla tacere, in particolare per i suoi coraggiosi reportage sulle violazioni dei diritti umani in Cecenia per responsabilità dell’esercito russo. Fu chiaramente un omicidio di Stato, con chiare e complicità del regime di Putin. Da allora Anna Politkovskaja è diventata un simbolo di libertà, come Dafne Caruana Galizia, Ilaria Alpi e Giulio Regeni. Regeni. L’altro ieri Putin ha concesso la grazia ad uno degli organizzatori di quell’omicidio e lo ha fatto perché quel detenuto quel detenuto aveva accettato di andare a combattere con l’esercito russo nella sporca guerra contro l’Ucraina. La grazia non era un atto dovuto: ai detenuti che hanno accettato di andare in Ucraina al massimo veniva ipotizzato un ricalcolo di pena. No, Putin gli ha concesso la grazia e questo è apparso quasi come un premio, certamente come un segnale di riconoscenza. E lo fa mentre sta assestando ulteriori strette a giornali, radio, TV, giornalisti e blogger. Dopo questo gravissimo atto, noi vogliamo anche in questa sede ricordare il sacrificio di Anna Politkovskaja, la cui memoria è stata di nuovo oltraggiata, come ha detto il il direttore di «Novaja Gazeta», il premio Nobel per la pace Dimitri Muratov. Lo vogliamo fare per lei, per la figlia Vera che tiene vivo l’impegno civile della madre e quello per la libertà di informazione. signora Presidente, nel 2007, dopo l’assassinio, il Comune di Roma le dedicò uno spazio, un bello spazio a Villa Pamphili. Vera, la figlia, era lì

è stato ospite Taghi Rahmani, giornalista, attivista iraniano, marito del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, rinchiusa nelle carceri del sanguinario regime iraniano. regime iraniano. Non dimentichiamo mai che i regimi uccidono, rinchiudono, fanno tacere le voci libere. Le democrazie difendono quelle voci, le libertà che hanno conquistato e devono farlo a partire da quelle dell’informazione e del giornalismo d’inchiesta. Le democrazie sono vicine alle troppe persone che, per praticare queste libertà, pagano anche con la vita, proprio come Anna Politkovskaja.

Signor Presidente, prendo la parola oggi, con ventiquattro ore di ritardo, perché per qualche motivo, inspiegabilmente, la Presidenza del Senato non mi ha dato la parola ieri, quando l’avevo richiesta. Avrei voluto parlare ieri per commentare e portare all’attenzione dell’Assemblea e del Paese che quest’Assemblea rappresenta la decisione della Corte suprema britannica, che ha dichiarato l’accordo intercorso tra il Governo di Rishi Sunak e di Suella Braverman e il Ruanda per il per il trasferimento coattivo dei migranti in Ruanda unlawful, che in inglese vuol dire illegale. Voglio commentare questa decisione della Corte suprema perché evidentemente quell’accordo è stato il modello assunto dalla presidente Meloni per la stipula dell’accordo con l’Albania, che nello stesso modo intende esternalizzare la gestione dei migranti presso un Paese terzo. Il ritardo dovuto al diniego della parola da parte del presidente La Russa, che mi costringe a parlare oggi, mi dà però anche l’occasione di commentare quello che ha detto la Commissione europea, che ha spiegato che questo accordo intanto sta in piedi in quanto è esterno al diritto dell’Unione e quindi si applicherà eventualmente soltanto ai salvataggi fatti in acque terze, quindi in acque internazionali. Tutto questo per dire che noi siamo in presenza di un accordo con l’Albania del quale questo Parlamento ancora non sa nulla. Le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana alla Camera dei deputati che il Governo venga urgentemente a riferire su questo accordo. Mi pare di capire che dalla Presidenza della Camera ci sia un’apertura in questo senso. Voglio quindi sollecitare anche la Presidenza del Senato far valere le prerogative di questa Camera che, come dicevo, rappresenta l’intero Paese, perché è un diritto del Paese sapere esattamente questo accordo cosa contiene, come si intende applicarlo, quali sono le risposte rispetto alle evidenti complessità umanitarie e organizzative. e organizzative. La mia richiesta è questa, segnalando che al primo test di prova di un accordo di questo genere un tribunale, sebbene straniero, ha già stabilito che questo tipo di accordi è all’esterno del diritto internazionale e umanitario.

per la mia generazione un esempio di donna impegnata nelle istituzioni e nella società per cambiare la vita delle altre donne, di tutte, scrivendo leggi adeguate a promuovere i loro diritti e la loro libertà. Era entrata nel Parlamento nel 1976, insieme a un’onda di giovani deputati che costituirono l’intergruppo delle donne comuniste, un’intuizione importante del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, portando in Parlamento lo sguardo e il punto di vista autonomo delle donne. Oggi a Messina la ricorderà Romana Bianchi, che dirigeva e coordinava quell’intergruppo. Angela Bottari era nata a Messina, si è impegnata anche nella sua città, prima come consigliera comunale e anche dopo la sua esperienza parlamentare come assessore. È davvero madre di leggi e di battaglie fondamentali per le donne di questo Paese. Fu la prima a scrivere una proposta di legge in cui la violenza sessuale diventava reato contro la persona e non contro la morale e fu la direttrice di quel testo, ma si dimise perché il dibattito parlamentare, all’epoca non ancora adeguato, aveva trasfigurato quella proposta. Ci vollero poi molti anni ancora

proprio come un’altra siciliana, Franca Viola, che nel 1965 si era rifiutata di accettare il matrimonio riparatore. Questo anche a sottolineare e a ricordare che le donne del Sud, fuori da ogni stereotipo, sono state un pezzo importantissimo della battaglia dei diritti delle donne di questo Paese. Angela Bottari fu anche impegnata contro la mafia. Legata profondamente a Pio La Torre, ricorda la sua partecipazione al comitato ristretto per la legge Rognoni-La Torre come una delle sue esperienze fondamentali di parlamentare. Lasciò, scelse di lasciare dopo tre legislature, ma si impegnò sempre nel partito, nel Comune, come ho ricordato, nella Fondazione Iotti, per cui ha curato anche per Donzelli una pubblicazione sul centenario di Nilde Iotti e anche del Partito Comunista, nella Conferenza delle democratiche. È lì che io l’ho incontrata, impegnata fino alla fine dalla parte delle donne e nel Partito Democratico. Per questo, per quello che è stata, per la sua passione, per le battaglie, per l’essere stata davvero una pioniera dentro le istituzioni, ci mancherà tantissimo.

(approvato dalla Camera dei deputati) (937) II. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione La seduta è tolta